Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, quando la Regione Campania presentò, a cavallo degli anni 1994-1995, il piano di smaltimento dei rifiuti...

era in carica il Governo Dini e dunque certamente non un Governo di centro-destra. Ebbene, bisogna chiedersi oggi perché quello che era considerato un ottimo piano da coloro che se ne intendono non ha funzionato ed è stato un totale fallimento. La prima considerazione da fare è la seguente: il piano in questione prevedeva per lo smaltimento dei rifiuti, al termine del ciclo, la realizzazione di due termovalorizzatori per bruciare il CDR e produrre energia.

grazie all'intervento dell'allora Ministro dell'interno che faceva accompagnare gli operai, le maestranze, che dovevano realizzarli dai carabinieri o dagli agenti di pubblica sicurezza. La seconda considerazione che voglio fare è che il commissariamento avvenne nella prima fase, non solo in Campania ma anche nelle altre Regioni, nominando commissari i prefetti: il fallimento fu totale. Chi governava allora pensò, dunque, di non rivolgersi più ad alti funzionari dello Stato, ma di commissariare ricorso alla politica, quindi con i presidenti delle Regioni o comunque con delegati dei presidenti delle Regioni. Anche in quel caso, il fallimento fu totale.

i cumuli di spazzatura arrivasse spesso anche ai primi piani. E se qualcosa deve essere rimproverato ai politici nazionali, è sicuramente il non essere stati capaci di convincere i cittadini in buona fede che la realizzazione dei termovalorizzatori era l'unico mezzo per poter risolvere il problema.

che vuole mantenere lo *status quo* perché mantenendolo continua ad arricchirsi, come ha fatto in questi ultimi dieci anni. C'è stata omertà da parte di alcuni cittadini? Io non generalizzo, ma certamente ci sono alcuni che hanno fatto finta di non vedere, di non sentire e soprattutto di non parlare. Il Il Consiglio dei ministri ha deciso di presentare questo decreto‑legge e di proporre al Parlamento la nomina, come commissario straordinario, del dottor Guido Bertolaso:

Ci aspettavamo, però, che all'interno del provvedimento si fosse deciso di mettere in condizione Guido Bertolaso di poter veramente intervenire,

che sanno che in questi ultimi dieci anni sono stati inviati verso la Campania centinaia di miliardi per lo smaltimento dei rifiuti e, non essendosi risolto il problema, si ricorre nuovamente ai cittadini per far pagare loro, attraverso la tariffa, lo smaltimento dei rifiuti. Ma questi cittadini campani quante volte devono pagarne lo smaltimento? *(Applausi dal Gruppo* *AN)*. Lo pagano attraverso le tasse e ora si trovano a pagarlo ulteriormente attraverso la tariffa.

lo smaltimento dei rifiuti in Campania, senza ricorrere al soccorso di altre Regioni o inviando i rifiuti verso la Germania, com'è accaduto più volte. Ma ci devono essere le risorse. Non è nemmeno concepibile - circola questa voce, voglio sperare che non sia vera - che si trovino le risorse fino al 31 dicembre, poi si farebbe approvare un ordine del giorno. Questo è assolutamente inaccettabile per il Gruppo di Alleanza Nazionale. Noi siamo disponibili ed abbiamo apprezzato la scelta di Bertolaso, perché con la Protezione civile si ha alle spalle una struttura molto forte; quindi, Bertolaso va benissimo, però

esponenti autorevoli del Governo; ci facciano sapere quanti soldi sono disposti a prevedere in questo decreto e, un secondo dopo, avranno l'approvazione del Gruppo di Alleanza Nazionale. Pregherei i colleghi di prendere posto, perché è difficile intervenire in una situazione del genere. È iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi senatori, sono napoletano e, come tale, avrei gradito parlare delle bellezze di Napoli, del suo mare, del suo bel clima, dei suoi castelli, delle sue biblioteche, della sua università, della sua storia millenaria e della sua civiltà. Invece, oggi si parla e si sente parlare di violenza, di camorra, di morti e, infine, di rifiuti, che ammorbano l'aria e costituiscono un pericolo per tutti gli abitanti di questa nobile città. Guardando la realtà, mi sento mortificato di dover parlare in quest'Aula e davanti a tutta la Nazione della grave quanto insostenibile condizione in cui versa oggi Napoli; e questo nonostante i miliardi che Regione, Province e Comuni campani hanno sperperato e non hanno saputo amministrare, con la conseguenza che non sono stati capaci di tutelare neppure la salute dei loro cittadini. Com'è possibile che l'ordinario prelievo dei rifiuti e il loro necessario trattamento sia stato normale nel corso degli anni, senza stati e momenti di emergenza? Com'è possibile che in 12 anni la situazione sia precipitata, passando via via nelle mani di diversi commissari straordinari, per giungere ora ad un risultato fallimentare, ad uno stadio di emergenza nazionale, tanto da dover ricorrere al capo del Dipartimento della protezione civile, dottor Bertolaso? Dopo tanto clamore e molteplici polemiche...

è stato ora emanato un ennesimo decreto, nato insufficiente, debole, senza coperture finanziarie e, in più, addirittura incostituzionale. Ora è il momento di fare sul serio e di arrivare ad un piano che liberi ed estirpi questo problema che affligge Napoli. Signori della maggioranza, il commissario Bertolaso vi ha avvertito: se il decreto‑legge in discussione in Parlamento non conterrà poteri e strumenti necessari per fare un buon lavoro, sarà costretto a dimettersi. Non è possibile che un commissario...

prego di prendere posto e di abbassare il volume della conversazione tra di voi, altrimenti è difficile parlare in questo contesto. Non è possibile che un commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania non abbia i poteri e gli strumenti idonei per risolvere il problema una volta e per sempre: Bertolaso ha detto apertamente che questa è l'emergenza più difficile che ha dovuto affrontare da quando ricopre la carica di commissario della Protezione Civile. Questo decreto, così come si prospetta, è quasi una camicia di forza che si vuole imporre al commissario Bertolaso senza dargli gli strumenti necessari per la soluzione del problema. Come ho già detto, c'é l'incapacità degli amministratori campani, di Regione, Provincia e Comuni, che non hanno saputo svolgere i loro compiti e oggi vogliono scaricare completamente sulla Protezione Civile questa loro responsabilità. È strano

richiami. Gli argomenti sono importanti: chi vuole parlare d'altro, può accomodarsi fuori, altrimenti è veramente impossibile governare l'Aula. Prego, senatore Pontone, le chiedo scusa a nome dei colleghi. fino ad aizzare la gente per impedirne la realizzazione, oggi che sono al Governo ne vogliano la costruzione. Signori della maggioranza, Napoli, la mia Napoli, sicuramente non può morire e non morrà per colpa vostra. ringrazio senatore Pontone, anche per le difficoltà nelle quali è intervenuto. È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha facoltà. Signor Presidente, ancora una volta quest'Aula si trova ad esaminare un provvedimento che riguarda l'emergenza rifiuti in Campania. Allora, una riflessione è doverosa per individuare le responsabilità che ci sono state in questa che è stata definita una vergogna altrimenti non acquisiremmo esperienza dal passato e non potremmo adottare gli opportuni provvedimenti. Ebbene, basta riguardare il piano così come era stato formato per individuare il il dilettantismo con il quale è stata affrontata la questione. Un sistema montuoso fatto di CDR, incapace anche di essere bruciato, senza pensare al termovalorizzatore, vale a dire alla fase finale necessaria per consumare tutto ciò che viene raccolto e viene prodotto. Ma, soprattutto, in questo periodo c'è stata un'inefficienza, un clientelismo, una scandalosa gestione del commissariato, che pure non è cosa nuova. Già nel 2001 la Corte dei conti l'aveva sottolineato con parole dure, con rilievi che erano indicativi di un certo tipo di gestione: in modo particolare, aveva sottolineato l'inefficienza organizzativa di quella gestione, con costi elevati e scarsa produttività complessiva,

del Ministero delle finanze; il dottor Natale Monsurrò ha sottolineato come la struttura addirittura operava senza un bilancio di previsione di entrata e di spesa e ha indicato anche alcuni casi veramente scandalosi: la costituzione della società PAN fatta insieme ad una società di informatica con 100 dipendenti, addirittura con compensi che fanno tremare le vene ai polsi, relativi alla costituzione di una società presieduta dal dottor Riccardo Di Palma, compensato con 400.000 euro senza che nulla avesse dimostrato di aver fatto in quel frattempo. Sono elementi che emergono da atti ufficiali, sui quali mai si è intervenuto e dei quali mai si è preso atto con responsabilità. Ma il fatto eclatante, signor Presidente, è la è la famosa assunzione nel 2001, vale a dire alla vigilia di un appuntamento elettorale, di ben 2.314 LSU a tempo indeterminato, per un costo di 55 milioni di euro annui.

quel fenomeno, ha avuto quella responsabilità così alta, ma anche nella relazione presentata dalla Commissione di indagine sui rifiuti, dove sono stati segnalati casi vergognosi: terreni che passano di mano in una sola giornata 4 a 5 persone, con un aumento di prezzi stipulati dalla stessa persona nei confronti della stessa società e presso lo stesso notaio. Pare vi siano ben 40 procedimenti penali e che 14 magistrati si interessino della vicenda. Ma

Proprio in questo momento, signor Presidente, è arrivato un comunicato stampa da parte del commissario Bertolaso che ha minacciato le proprie dimissioni, denunziando in maniera chiara e precisa le responsabilità degli enti locali, che sinora nulla hanno fatto verso questo fenomeno. Inoltre, è stato fatto un paragone

nei confronti di questa emergenza, anche lo stesso Bertolaso si dichiara impotente ed incapace di potere intervenire con efficacia e con efficienza. Quali i rimedi? Innanzitutto, la individuazione della responsabilità di coloro i quali volevano contrabbandarci un drammatico quanto ridicolo Rinascimento e la voglia forte di tornare ad una normalità per cancellare quella che è stata giustamente definita una vergogna nazionale. Quali i criteri? Lo abbiamo detto e più volte sottolineato. Innanzitutto, la provincializzazione dei rifiuti: ciascuna Provincia deve raccogliere e smaltire i rifiuti che produce. Soprattutto si sente la necessità di una responsabilizzazione e di un coinvolgimento degli enti locali, in modo particolare dei Comuni e delle Province che sinora si sono sottratti a quel compito, anche se indotti da una gestione

nell'esprimere il voto sul mandato al relatore, ha espresso un voto di astensione per alcuni motivi che succintamente riepilogo: alcuni sono stati illustrati dai colleghi intervenuti durante la discussione generale e riflettono le responsabilità di una vicenda assai triste per l'intera Nazione, quale quella dell'emergenza rifiuti in Campania. Condivido interamente il contenuto dell'intervento dei colleghi

A lume delle mie conoscenze, signor Presidente, onorevoli colleghi (mi spiace che in questo momento molti senatori siano impegnati in conciliaboli vari), non esiste una tariffa regionale di smaltimento dei rifiuti.

dell'articolo 5 del decreto-legge in esame, poi ripreso da un emendamento della Commissione elaborato sul testo definito dalla 5a Commissione permanente, sottintendesse la volontà una nuova forma di tariffazione dello smaltimento dei rifiuti effettuata su base regionale. Ciò sarebbe, innanzi tutto, un'innovazione ed un ulteriore aggravio, cioè l'introduzione di una nuova forma di aggravio nei confronti dei cittadini,

alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Quindi, il Governo e la 5a Commissione permanente devono rassicurarci sul significato della dizione "tariffa di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania":

e contrari ad ogni forma, anche surrettizia, di introduzione di nuove tassazioni e vessazioni del cittadino campano, che è già sufficientemente provato dall'inefficienza dei servizi locali che hanno provveduto al servizio di smaltimento dei

prego di fare silenzio. Chiunque voglia parlare si può accomodare fuori dall'emiciclo e dall'Aula, altrimenti è difficile sviluppare un intervento.

di conseguenza, il Governo ha l'obbligo di indicare le risorse che metterà a disposizione del commissario straordinario da oggi a quella data. Tali risorse sono facilmente quantificabili, anche sulla base delle esperienze precedenti (per quanto queste non abbiano portato a soluzione definitiva del problema). Il Governo Berlusconi, per un analogo periodo di tempo, ha messo a disposizione del commissario straordinario 80 milioni di euro. Richiediamo

che valuteremo l'atteggiamento da assumere su questo decreto al termine della discussione sugli emendamenti e quando il Governo avrà fornito i chiarimenti da noi richiesti. Signor Presidente, signori senatori, nel motivare il voto favorevole del Gruppo dell'Ulivo alla conversione in legge la franchezza mi obbliga a non tacere il senso di sproporzione che si avverte dalla lettura del provvedimento. Tra il provvedimento e la gravità della situazione che si cerca di fronteggiare c'è una sproporzione che si può leggere già nel titolo, nel senso che il ricorso alla decretazione è giustificato in nome dell'emergenza ma il contenuto del decreto non basta affatto ad uscirne. Ciò non vale solo per la copertura dei costi, che la tariffa regionale non basterebbe sicuramente a compensare, e che ora vedo da un emendamento della Commissione sarà affidata ai fondi di dotazione del commissario, ma per considerazioni più ampie che cercherò di presentare in breve. La necessità del decreto è fuori discussione e non manca neppure qualche elemento di utilità di cui vorrei parlare fra poco. In premessa, dopo gli esiti infausti delle precedenti gestioni commissariali è senz'altro utile la chiamata in campo del Servizio nazionale di protezione civile e la nomina a commissario del capo del servizio Guido Bertolaso, funzionario che ha dimostrato nelle circostanze più difficili la capacità di servire lo Stato e i cittadini nelle operazioni di prima linea. Mi sembra che su questo siamo tutti d'accordo. Tanto basta di fronte alla somma urgenza delle cose per votare la conversione in legge del decreto ma con l'amara cognizione che ciò non basterà affatto ad uscire dall'emergenza. Signor Presidente, fra le anomalie del caso italiano ci sono gli ossimori delle emergenze eterne. Quella dei rifiuti in Campania decorre ufficialmente dal 1994, come ci ha ricordato stamane il relatore, ed è appunto un'emergenza eterna di strade ingombre di rifiuti fino al rischio per la salute pubblica, in un'area fra le più sovraffollate di Europa e fra le poche d'Italia ad alta densità di popolazione infantile. Un'emergenza eterna di discariche, per lo più fuori norma, dove razzola di tutto, soprattutto la malavita. Un'emergenza eterna di termovalorizzatori, localizzati progettati e non costruiti, e di rivolte popolari che occupano strade e ferrovie per protestare non contro i cumuli di immondizie, ma contro gli impianti che sarebbero necessari per rimuoverli. Posso rivendicare qualche precedente in proposito soltanto per ammettere una sconfitta. Anni fa provai ad occuparmi, quale privato cittadino del Nord, del degrado ambientale dei Campi Flegrei e del litorale domiziano, un patrimonio storico, culturale e naturale unico al mondo, tappa obbligata del *grand tour* italiano dei viaggiatori europei del Settecento, che versava - l'uso del tempo passato è sbagliato per ottimismo - in condizioni tali di dissesto ecologico già negli anni Ottanta, quando mi riuscì di firmare la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, a individuare la zona flegrea e il basso Volturno come una delle aree a più alto rischio ecologico cui applicare le misure straordinarie istituite da quella legge. Quando qualche anno fa tornai ad occuparmene, due parlamentari napoletani - l'onorevole Gerardo Bianco, alla Camera e il professor Fulvio Tessitore, qui al Senato - se ne fecero portavoce con un allarmato articolo sul quotidiano «Il Mattino». Sono passati altri tre o quattro anni e la questione rimane agli onori delle cronache non solo italiane, ma internazionali. La stampa estera commenta con sarcasmo le spedizioni ferroviarie dei rifiuti napoletani in varie parti d'Italia e d'Europa al non modico costo - si legge adesso nella relazione al decreto - di 140 euro per tonnellata. La Campania produce circa 7.200 tonnellate di rifiuti al giorno: uno spreco enorme di denaro pubblico, un'enorme assurdità ecologica. È perciò desolante, anche se a breve inevitabile, leggere nel decreto la previsione secondo cui una parte non precisata dei rifiuti prodotti in Campania continuerà ad essere trasferita fuori Regione. una parte che non viene precisata perché per trasferirli tutti si spenderebbe, come si è visto, la bellezza di un milione al giorno. Quale contributo porta dunque il decreto, che indichi almeno un percorso per venire fuori dall'eterna emergenza? A mio avviso il solo efficace, oltre agli interventi immediati di somma urgenza, è l'insieme di misure per la raccolta differenziata, che in Campania segna, sia pure con qualche eccezione meritoria, indici fra i più bassi in Italia: poco più del 10 per cento rispetto alla soglia di norma del 35. Sul punto, in effetti, nel decreto qualcosa di utile c'è: c'è la nomina di un subcommissario con l'incarico specifico di promuovere e coordinare la raccolta differenziata; c'è la possibilità di nominare commissari *ad acta* nei Comuni inadempienti; e, soprattutto, è sperabile che si applichi alle campagne per la raccolta differenziata l'articolo 2 del decreto, che dispone il programma di informazione e partecipazione dei cittadini, perché la raccolta differenziata, che è la prima misura fondamentale per una gestione razionale del ciclo, dipende tutta dal civismo della popolazione e quindi richiede davvero una campagna di educazione ambientale nelle scuole, nelle associazioni locali, nelle comunità di vicinato. Se questo è l'elemento del decreto più promettente per uscire dall'emergenza, il limite più grave consiste, a mio avviso, nel silenzio sulla chiusura del ciclo, ossia sull'individuazione definitiva dei siti e delle costruzioni di impianti per il recupero energetico dei rifiuti non riciclabili. Il decreto non dice nulla in proposito, ma dalle notizie che circolano - perché si sa o si pensa di sapere - è emerso che dei siti a suo tempo individuati non ne sopravvivano ormai più di un paio che dei termovalorizzatori in costruzione ve ne sia soltanto uno, che sarà idoneo a bruciare in un anno 650.000 tonnellate di rifiuti, quanta la Campania ne produce in meno di tre mesi, nel casertano, pare che i macchinari siano stati acquistati da anni e restino nei depositi dei venditori in attesa di costruzione dell'impianto. Quindi, di fronte allo spreco finanziario della spedizione fuori Regione e all'assoluta insufficienza degli impianti di incenerimento, anche nel futuro di medio termine, il decreto ripiega sulla riapertura delle discariche che - si legge nella relazione, con riferimento all'articolo 5 - «allo stato attuale, rappresentano l'unica valida soluzione in grado di superare temporaneamente la fase di vera e propria emergenza ambientale». Le discariche della Campania sono oggetto di decine di provvedimenti giudiziari di validità ambientale quantomeno discutibile, mentre indiscutibile è purtroppo la connessione fra i depositi illegali in discariche non controllate e i profitti della camorra. A questo riguardo, un elemento utile viene non dal decreto, ma dal patto per la sicurezza di Napoli e Provincia, che dovrebbe essere sottoscritto - credo oggi o domani - dal Governo e dai poteri locali: il patto aumenta di trenta unità l'organico del reparto territoriale dei Carabinieri di Castello di Cisterna e aggiunge altri venti carabinieri al nucleo operativo ecologico per contribuire alle indagini oggetto di annose inchieste parlamentari mai concluse. Chi, come me, voterà per la conversione in legge del decreto non può certamente illudersi che questo basti ad uscire dall'emergenza eterna e ad avviare la gestione del ciclo dei rifiuti in Campania verso la normalità: ci si arriverà soltanto quando si riuscirà ad affermare un principio elementare di gestione ecologica talmente semplice che non occorre, per motivarlo, scomodare scomodare i sommi princìpi di sostenibilità affermati nella Carta di Aalborg, cui fa appello l'articolo 2 del decreto. Non occorre essere degli specialisti in materia di sostenibilità ambientale per rendersi conto che ogni territorio deve farsi carico di smaltire i rifiuti che produce, anziché accatastarli in balle plastificate sui frutteti di Aversa, in attesa di spedirli per ferrovia. C'è in gestazione da anni una legge regionale in materia; c'è o c'era il piano dei termovalorizzatori, che funzionano egregiamente in tutta Europa e che non possono essere oggetto di anatema in nome della sindrome Nimby che, in questo caso, non serve neppure a proteggere il cortile di casa; e, sugli illeciti, c'è la *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre (ho concluso Presidente), che ha pubblicato la legge istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta, erede anche quella di emergenze su cui si indaga fin dalla XII legislatura. È lecito attendere che l'inchiesta parlamentare faccia pulizia nella materia ed io mi permetto di dire, concludendo, che lo scandalo civile e lo spreco finanziario non possono durare oltre, per non offendere oltre una città nobilissima ed una Regione che, nonostante i guasti cui è sottoposta, appartiene al patrimonio ambientale dell'umanità.

Il collega D'Alì e, prima di lui, il collega Matteoli sollevavano il problema delle risorse disponibili che accompagnano questo provvedimento e richiamavano, in particolare, una critica a una tariffa di smaltimento di rifiuti di tipo regionale. Credo che questa interpretazione derivi da una formulazione non adeguata del testo

perché c'è un'attività ordinaria di gestione dei rifiuti in Campania che interferisce con l'attività del commissario, quindi i proventi della TARSU vanno citati, in quanto fanno parte delle misure necessarie e in atto. Si aggiunge, nell'emendamento 5.100, approvato dalla Commissione: «nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato». Come i colleghi già sanno, in Commissione, il Governo ha individuato una disponibilità finanziaria che riguarderebbe questi due mesi del 2006; la difficoltà contabile è impegnare risorse sull'esercizio 2007 mentre è in corso la sessione di bilancio. però, che l'impegno politico, che potrebbe essere formalizzato dall'Aula, è di coprire questi due mesi grosso modo secondo la cadenza delle quote individuate anche dall'opposizione e poi impegnarsi, per la parte restante, ad individuare le risorse nell'ambito dei fondi della Protezione civile per le emergenze straordinarie, risorse che ci sono e che vanno

grosso modo nella misura in cui veniva stimata, cioè in circa 80 milioni di euro. Ripeto: il problema è che noi non siamo in grado. Credo sia così, a meno che qualcuno non riesca a trovare una soluzione. Siamo in grado di coprire due mesi a chiusura dell'esercizio 2006,

alla loro approvazione) vadano nella direzione di fornire strumenti, risorse e tempi certi rispetto alla fuoriuscita dalla gestione commissariale e soprattutto

campano: il problema dell'emergenza campana è ormai un'emergenza nazionale. È con questo spirito che dobbiamo affrontare il prosieguo della discussione in quest'Aula.

sul decreto-legge relativo all'emergenza nel settore rifiuti in Campania, partendo innanzitutto dalla necessità di dare atto a tutti i Gruppi della maggioranza e dell'opposizione dell'atteggiamento costruttivo di cui hanno dato finora prova per consentire l'*iter* parlamentare del decreto e il suo approdo in Aula nei termini fissati dal calendario dell'Assemblea e della disponibilità che si è appalesata, nonostante qualche elemento di criticità, emerso nel dibattito, relativo soprattutto al rapporto tra le necessità finanziarie che un'emergenza quale quella dei rifiuti nella Regione Campania manifesta e le disponibilità che è possibile assicurare a sostegno dell'azione del commissario. Desidero soltanto ricordare, come hanno già fatto tutti i senatori intervenuti, che questo decreto si colloca a dodici anni

più forte delle precedenti, decidendo di nominare commissario per l'emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile. Sono lieto che questa decisione del Governo (che è un po' il cardine del decreto perché poi su questa scelta è costruito l'impianto del decreto sia stata salutata con favore da tutti i rappresentanti dei Gruppi intervenuti nel dibattito, oltre che dall'opinione pubblica, non solo perché la persona scelta ha dato buona, anzi ottima prova di sé in tante circostanze e di fronte a tante emergenze nelle quali il Paese si è imbattuto, ma soprattutto perché la formula di collegare l'intervento del commissario alla struttura e alle risorse ordinariamente a disposizione della Protezione civile ci pone nella condizione di rendere comunque più efficace l'azione del commissario

allo smaltimento, dal trasporto, alla destinazione finale dei rifiuti. È tutto il ciclo dei rifiuti che è chiamato in causa in questa emergenza della Campania e che richiede un intervento forte da parte del commissario, ma anche, probabilmente, dei raccordi con la politica ordinaria in materia, che bisogna assolutamente evidenziare nella prospettiva, peraltro, di una conclusione, rapida, nei limiti del possibile, della gestione commissariale. Non c'è dubbio che una gestione commissariale così lunga descrive una situazione patologica, non esprime una situazione fisiologica. Noi dobbiamo riuscire a far sì che questa patologia, anche se ha dei segnali, delle caratteristiche di cronicità, non assuma segnali di incurabilità. Ecco la ragione per la quale noi pensiamo - ci siamo trovati tutti d'accordo nel dibattito in Commissione, oltre che in Aula - di dover raccordare le azioni straordinarie e di emergenza che il commissario deve compiere all'ordinario che si deve poter svolgere con l'aiuto, con la collaborazione, con il protagonismo diretto soprattutto degli enti locali, della Regione, dei Comuni, delle Province, che agiscono anche attraverso i consorzi, ma anche dei cittadini. Il collega Ronchi sa,

da parte di tutti coloro che producono e smaltiscono rifiuti. Gli elementi di criticità emersi sono stati corretti da numerosi emendamenti della Commissione ambiente, che nell'insieme hanno sicuramente migliorato il testo, anche sulla base di osservazioni pervenute dalla Commissione affari costituzionali e di osservazioni e condizioni pervenute dalla Commissione bilancio.

a prevedere l'utilizzazione di risorse indirette (ricordo che la Ragioneria, fino ad ora, aveva previsto come copertura del decreto uno schema di copertura

ulteriore corrispondente impegno per far fronte alla prosecuzione del mandato del commissario che abbiamo tutti insieme convenuto debba finire il 31 dicembre 2007, noi ci auguriamo a completo superamento

che sono stati assunti in Commissione e che si assumono questa sera in quest'Aula.

la possibilità di coinvolgere le amministrazioni pubbliche e le strutture del Servizio nazionale della protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 1, rientra già nella competenza ordinaria del Capo del Dipartimento della protezione civile, che riveste anche il ruolo di Commissario delegato; le misure volte all'informazione e alla partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 2, rientrano tra le competenze ordinarie ed istituzionali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui il Dipartimento della protezione civile già fornisce supporto e collaborazione; rilevando tuttavia l'opportunità, al fine di garantire l'effettiva invarianza finanziaria del provvedimento, di riformulare il disposto normativo in coerenza con quanto rappresentato nella relazione tecnica e nei chiarimenti del Governo in merito alle modalità di copertura del provvedimento, precisando espressamente: - in relazione all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che la riduzione dell'organico della struttura commissariale di cui al comma 4 deve riferirsi a posizioni effettivamente occupate e risultare contestuale ed equivalente finanziariamente alla nomina dei sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al comma 3; che le attività di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 1, devono comunque essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; - con riferimento all'articolo 4, che i relativi oneri sono a carico del Commissario delegato, nel limite delle risorse a tal fine disponibili; che gli oneri derivanti dagli interventi per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonché quelli per la bonifica, messa in sicurezza e apertura delle discariche di cui all'articolo 5, sono posti a carico delle risorse rivenienti rivenienti dalla tariffa di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania, nonché degli ulteriori fondi disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 2, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; *b*) che al comma 4 del medesimo articolo 1, sia soppressa la parola: «successive» e che siano aggiunte, in fine, le seguenti: contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; che all'articolo 2, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; *d*) che all'articolo 4, dopo il comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente: Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Commissario delegato, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili.»; *e*) che all'articolo 5, il comma 6 sia sostituito dal seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza e apertura delle discariche di cui al presente articolo 5, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania, nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato».

1.11, 3.1, 1.13, 3.2, 5.0.2, 4.3, 5.1, 5.300, 5.7, 5.11, 5.26, 5.0.1, 6.2 e 7.20, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 5.9, sulla quale il parere è contrario. Formula infine parere non ostativo sui seguenti emendamenti, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'emendamento 1.14, dopo le parole: «di due terzi» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; all'emendamento x1.0.1, al comma 1 del capoverso «Art. 1-*bis*», dopo le parole: «ad adottare,» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»; all'emendamento 2.1, dopo le parole: «Il Commissario delegato» siano inserite le seguenti: «,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»; *d*) all'emendamento 4.7, dopo le parole: «I commissari *ad* *acta* definiscono,» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

sia sostituita dalla seguente: «devono», nonché parere di nulla osta sull'emendamento 4.200, condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, alla sostituzione, al comma 6, della parola: «possono» con la seguente: «devono». Esprime, poi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 3.300/6, 5.120/1, 5.120/2 e 5.100/1, e parere di nulla osta sul subemendamento 4.200/1, a condizione che, ai sensi della citata norma costituzionale, dopo le parole: «I commissari *ad* *acta* definiscono,» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti esaminati».

bisognerebbe che io avessi il tempo di riunire almeno il Comitato pareri, perchè è un emendamento che ha un rilievo finanziario piuttosto significativo, per cui non posso dare il parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento. PRESIDENTE. Senatore Morando, l'emendamento è già stato trasmesso alla Commissione

che mi sembra giusto prevedere, che la gestione commissariale possa finire prima nel caso in cui, ci auguriamo, finisca prima l'emergenza. In secondo luogo, ho parlato di coinvolgimento degli enti locali:

degli emendamenti della Commissione. Perché queste due questioni? Perché, come si è visto anche dal dibattito,

perché nel contenuto di questo emendamento vi è in effetti la motivazione vera della crisi che ha attanagliato la nostra Regione. Dico questo perché lo scollamento che si è creato tra le Province e la Regione è così forte che, se non lo si supera

vada sul territorio e si trovi di fronte una situazione di questo tipo difficilmente riuscirà a risolvere i problemi. I presidenti delle Province, che si sono visti esclusi (mi riferisco alla fase 1999-2004, quando la carica di commissario straordinario coincideva con quella di presidente della Regione Campania), rimproverano al presidente rimproverano al presidente della Regione di aver agito in perfetta solitudine e di aver utilizzato le risorse senza un minimo di razionalità. Io penso che, se coinvolgiamo le Province in un ragionamento, in un discorso, in un percorso di operoso dialogo, possiamo immaginare di poter risolvere il problema. Ecco perché ho ritenuto di presentare l'emendamento 1.11. Per quanto riguarda l'emendamento 1.13,

è coadiuvato da una commissione o da più comitati tecnici. Io mi sono permesso di individuare, attraverso questo emendamento, i soggetti istituzionali che sono tenuti a dare una specifica collaborazione: il CONAI, l'ARPAC, l'APAT e altri organismi. Penso che, con questo emendamento, possiamo

tutti i colleghi che sono intervenuti - il decreto è privo di copertura finanziaria; è arrivata una timida disponibilità per uno o per due mesi. Ma noi dobbiamo dare un segnale di cambiamento: o in Campania si volta pagina e si fa sul serio, oppure ciascuno si assume le proprie responsabilità, e allora non serve il decreto, non serve il commissario, ognuno faccia la propria parte.

seduta per qualche minuto per attendere l'arrivo del senatore Morando con il parere sull'emendamento

a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 6, le parole: ", che viene a tal fine integrata dell'importo" siano sostituite dalle seguenti: Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilità della citata contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l'importo"».

la Commissione ed il relatore accettassero una modifica del testo. Forse per l'economia dei nostri lavori, al fine anche di consentire alla Commissione bilancio di considerare chiusa la questione, bisognerebbe vedere se il relatore è

sulla procedura. In particolare, vorrei sapere se in questo caso si applica il comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento, ovvero se lei mette in votazione la richiesta di votare per parti separate.

*(FI)*. Il Gruppo di Forza Italia voterà in maniera particolarmente convinta la modifica al comma 3 che prevede la sostituzione della previsione di tre subcommissari con quella di un subcommissario. Abbiamo fatto i salti mortali per cercare di reperire le somme. Sarebbe bene che il decreto fosse virtuoso dal punto di vista dell'economia in tutte le sue parti, anche se questa certamente non è estremamente rilevante ai fini della spesa complessiva. Questa previsione di tre subcommissari a noi non convince, preferiamo che ce ne sia uno solo e con poteri vicari, il che comporterebbe sicuramente un'economia e anche una migliore identificazione del quadro di riferimento operativo. questa proposta di modifica al comma 3 e spero che anche i colleghi della maggioranza si convincano della bontà di questa proposta.

**Il Senato non approva.** Senatore Matteoli, c'è un invito al ritiro dell'emendamento 1.1 da parte del relatore, lo accoglie?

Dichiaro aperta la votazione. Colleghi, seduti per cortesia.

alla destra della senatrice Procaccini. Se è sparita la tessera, veramente apro un'indagine con perquisizione.

ed esprimono pareri che sono molte volte espressi da enti istituzionali. Ebbene, questo emendamento non fa altro che radunare tutti gli enti che in materia hanno una competenza specifica e che pertanto potrebbero dare

agli enti locali eletti, perché dopo 12 anni di commissari e di prefetti siamo ora arrivati al commissario ministeriale. Non vorrei che la prossima volta (visto il sicuro insuccesso che, suo malgrado

Credo che l'emendamento 1.15 corrisponda ai sentimenti espressi da tutti i Gruppi durante il dibattito in Commissione: la volontà di uscire fuori della gestione commissariale non può che tradursi in una disposizione normativa di tassativo ritorno alla gestione affidata agli enti territoriali.

una gestione a tempo il più limitato possibile. È giusto che gli enti locali si assumano la propria responsabilità verso i cittadini nella gestione di questo tema caldissimo.

la volontà condivisa è di arrivare entro il 31 dicembre del 2007 alla fine della gestione commissariale. Dirlo oggi, a fronte della situazione di emergenza che tutti i colleghi, anche dell'opposizione, hanno evidenziato, mi sembra

voglia evidenziare l'importanza della raccolta differenziata. Credo che anche i colleghi di Governo e i colleghi di maggioranza

Presidente, se non ho capito male, il Presidente della Commissione, nonché relatore, ha espresso parere contrario

ha chiesto all'Aula di votare a favore di un emendamento che, in qualche modo, sostiene la raccolta differenziata. Stento a credere che i colleghi della maggioranza, che hanno fatto più volte grandi polemiche perché il precedente Governo non aveva sufficientemente spinto verso la raccolta differenziata, si trovino ora a votare contro. Mi sembra un controsenso: sufficiente chiarimento su cosa si vota o evidentemente il relatore, nonché Presidente della Commissione, ha interpretato male un emendamento che a me pareva molto, molto chiaro.

perché se fosse vero il problema dell'assenza di copertura finanziaria bisognerebbe incrociare l'articolo 2 con il parere espresso dalla Commissione bilancio. Nel parere, tra l'altro nella premessa, cosa credo irrituale, la Commissione bilancio dice che «(...) le misure volte alla informazione e alla partecipazione dei cittadini, ai sensi articolo 2, rientrano tra le competenze ordinarie ed istituzionali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui il Dipartimento della protezione civile già fornisce supporto e collaborazione». La Commissione bilancio, cioè, dice giustamente che la campagna per la promozione della raccolta differenziata si può fare, ma la Protezione civile faccia riferimento alla Presidenza del Consiglio e quindi alle risorse della Presidenza del Consiglio e non quindi alle risorse previste

finanziaria, e cioè senza oneri aggiuntivi: si tratta di una previsione importante che segna davvero la volontà di fare la campagna di promozione. In caso contrario, francamente, stiamo discutendo del formalismo e non della sostanza delle iniziative che si intendono assumere.

**Il Senato non approva.**

Mi auguro che i Gruppi che ancora non lo hanno fatto, e sono pochi, trasmettano al più presto i nominativi per l'assegnazione dei posti, dopodiché si vedrà immediatamente chi si dedica alla musica durante le ore d'Aula.

Dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato non approva.**

Dichiaro chiusa la votazione.

Dichiaro aperta la votazione.

Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia nell'emendamento 2.30/6, che mi sembra assolutamente in linea con la Costituzione. Alla consulta regionale devono partecipare personalmente i sindaci, non i loro rappresentanti. Finiamola con questo giochetto della delega continua dei sub-commissari e dei rappresentanti; ognuno si assuma la propria responsabilità. Alla Consulta regionale devono partecipare i sindaci, non i loro rappresentanti, che non sappiamo oggi chi siano.

che non consente a noi un minimo di possibilità di trattativa. Questo decreto è entrato nelle Aule parlamentari

che c'è una rigidità a non far passare nemmeno un emendamento presentato dall'opposizione; ciò incattivisce l'Aula in un modo assolutamente inadeguato rispetto al provvedimento che andiamo ad approvare. FI).* È un provvedimento che non riguarda solo la maggioranza, ma riguarda tutti. Noi vorremmo contribuire a farlo passare, perché non abbiamo nessuna voglia di votare contro. Vediamo però, da un atteggiamento ostile,

Credo si sia creato un equivoco rispetto all'emendamento, da cui si è generata una forma ostruzionistica da parte dei colleghi della Lega. Mi riferisco all'emendamento 2.1, che avevo invitato il senatore Stefani e Leoni a

3.1, abbiamo ampiamente illustrato all'Aula che i dodici anni di gestione commissariale sono stati caratterizzati da notevoli sperperi.

Presidente, l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Coronella mi pare di buon senso e deriva anche dell'esperienza maturata sul territorio: chi segue e ha seguito le vicende dello smaltimento dei rifiuti e dell'emergenza in Campania sa benissimo che la maggior parte dei giudizi, delle controversie e delle consulenze sono state affidate a studi ben orientati. Ebbene la spesa, almeno per le notizie che siamo riusciti a recepire, solamente per consulenze è stata per uno studio napoletano di 16 milioni di euro. Non trovo nessun motivo per osteggiare questo emendamento posto che, nel momento in cui si vanno a ridefinire le condizioni per l'affidamento dei servizi di smaltimento, si chieda l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, Stato, un'avvocatura eccellente, fatta di professionisti che ben conoscono le questioni, specie quella campana, e che potrebbero dare la loro opera in maniera gratuita e secondo le proprie funzioni. Quindi, invito tutti a riflettere e ad evitare quello che appare un ulteriore sperpero di denaro.

3

**Il Senato non approva.**

Carrara, altrimenti qui non ci regoliamo. Poi, per quanto riguarda la Presidenza dell'Aula, capisco la sua stanchezza. Prima c'era il senatore Baccini, ora c'è lei: ma non c'è mai una turnazione?

Senatore Garraffa, mi sembra di aver dimostrato che tutte le richieste di intervento sono state osservate. osservate. Senatore Garraffa, dopo giustifico il senatore Storace quando si preoccupa per la mia

Fate a caso, per me è indifferente quale volete togliere. Siete quattro e ci sono cinque voti. Forza colleghi, l'abbiamo tolta? Una è di troppo.

nella quarta fila del secondo settore c'è una signora con i baffi, un signore con i baffi, che molto spesso urla

per evitare che si crei anche disinformazione rispetto all'esterno. La Commissione ha lavorato e ha prodotto questo emendamento che promuove fortemente la raccolta differenziata con obiettivi elevati del 35 per cento per i rifiuti urbani

si prevede al comma 3 e al comma 4 un impegno del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), che è inadempiente per molti versi, soprattutto nel Mezzogiorno, oltre a campagne informative.

cui il territorio è già stato gravemente colpito. Con questo articolo diamo anche la possibilità di aumentare le volumetrie disponibili delle discariche. Ricordiamoci la vicenda di Ariano Irpino, ricordiamoci la vicenda di Paenzano 2, discariche che hanno subito anche provvedimenti giudiziari tutt'ora in corso. Noi chiediamo che in queste realtà non si possa assolutamente intervenire e permettere di aumentare le volumetrie disponibili. C'è un altro passaggio che ritengo importante, che riguarda la tariffa; il il Governo ha predisposto un ordine del giorno per la copertura dei costi di questo provvedimento che, secondo noi,

che è riconosciuta unanimemente, nessuno può negare che sia vero; una gestione che rischia di scaricare le proprie inefficienze ancora sulla tariffa, dunque sulle tasche dei cittadini, e badiamo bene, sulle tasche di quei cittadini che la tariffa o la tassa sui rifiuti l'hanno già pagata e non si sono visti

recuperati all'interno del bilancio della Regione Campania, un bilancio che - voglio evitare ogni polemica - è sotto gli occhi di tutti, un bilancio che viene utilizzato molte volte

andrebbero calibrati meglio: in periodi normali non meraviglierebbero più di tanto, ma mi pare che chi amministra questa Regione si dimentichi da troppo tempo di amministrare una Regione che viaggia in emergenza. Come ho già detto oggi, se ne deve ricordare

il riferimento alla possibilità del commissario di determinare l'aumento delle volumetrie disponibili in materia di interventi di sistemazione delle discariche, perché mi sembra un riferimento eccessivamente generico generico che renderebbe possibile anche un ampliamento a dismisura di tali discariche. Mi pare sia opportuno invece individuare un parametro certo che fissi un limite nell'esercizio di questa facoltà discrezionale del commissario. Non avendo ravvisato

che oltre ad essere Presidente della Commissione ambiente è anche campano, conosce molto meglio di me la situazione drammatica in cui versano alcuni territori e Comuni della Regione, i quali hanno pagato e pagano tutt'ora un prezzo altissimo in termini di danni ambientali, sociali, economici e alla salute dei cittadini. Sono quei territori nei quali sono stati prevalentemente ubicati discariche, siti di stoccaggio impianti per il trattamento di rifiuti: posso qui citare l'area nolana e del giuglianese. Se scorriamo l'elenco dei siti individuati, vediamo che a Giugliano è previsto un impianto di CDR,

Per tali ragioni, abbiamo chiesto di prevedere che il commissario delegato, nell'aprire nuovi impianti, non possa individuare ulteriori siti nei suddetti territori e Comuni. Mi è stata mossa l'obiezione, signor Presidente, che non sarebbe

che tali localizzazioni sono avvenute senza alcun criterio razionale, al di fuori di un piano organico che riguardasse la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania. Pertanto, propongo - se possibile

valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in Comuni diversi da quelli in cui sono stati già realizzati impianti durante la gestione commissariale dell'emergenza rifiuti». Non si fissa un divieto assoluto, ma si indica un criterio che deve presiedere all'esercizio di questa attività discrezionale del commissario delegato.

intervengo per illustrare l'emendamento 5.100/1 che porta la firma di tutti i Capigruppo in Commissione ambiente della Casa delle Libertà.

sono già penalizzati da una dissennata gestione del comparto rifiuti in Campania. Occorre che il Governo, come abbiamo chiesto, stanzi in maniera inequivocabile le somme necessarie all'attività del commissario (che noi stimiamo in un minimo di 80 milioni), così come nel precedente periodo di commissariamento era stato fatto dal Governo centrale.

e poi gli altri che sono qui davanti, nell'emiciclo, e che amabilmente continuano a chiacchierare, di prendere posto oppure di accomodarsi fuori dall'Aula. esempio, il senatore Montino, insieme ad altri colleghi, di consentire a chi deve intervenire di farlo in un modo decoroso.

Chi conosce le vicende di Difesa Grande, la discarica di Ariano Irpino - fra questi c'è sicuramente il relatore -, sa bene che quella discarica, pur situata in un agro di Ariano Irpino,

Perché questa particolare predisposizione dei commissari ad ubicare discariche in Campania al confine con il territorio pugliese? Una motivazione c'è, perché in questo caso tutti i commissari hanno avuto vita più facile nel governare il dissenso e la protesta sociale. Infatti questo non ha riguardato e non riguarda solo Difesa Grande per chi, come il relatore ed il rappresentante del Governo,

modo, chi conosce queste vicende sa che la discarica di Difesa Grande, chiusa e riaperta a fasi alterne, è stata ultimamente sequestrata per disastro ambientale. La domanda che pongo

Il Parlamento ha la capacità di bloccare i disastri ambientali al confine con un territorio che non è quello campano? Penso proprio di no.

vorrei porre una domanda in caso di parere negativo. La Commissione bene ha fatto quando, intervenendo sul comma 3 dell'articolo in riferimento ai rifiuti trasferiti in altre Regioni, laddove si chiedeva l'ascolto dei Presidenti delle altre Regioni, ha trasformato tale ascolto in un'imposizione di concerto.

l'impatto ambientale e l'impatto socio-economico e produttivo, in questo caso non si chiede niente, non si concerta. È più importante il luogo materiale dove si va a depositare il rifiuto o sono più importanti gli effetti che da tali rifiuti derivano? Se sono, come sono, più importanti gli effetti, penso che quando si va a realizzare una discarica sull'uscio di casa altrui si ha il dovere di chiederne il concerto.

dovrà tener conto del carico ambientale e dei disastri ambientali provocati dalle discariche o da altri impianti già esistenti e in evidente stato di saturazione». Consegno alla Presidenza copia della

Barbato vada considerata insieme a quella del senatore Palumbo, che proponeva una formulazione che integrasse le due. Sarei dunque disposto ad esprimere un parere favorevole, modificando però

dalle discariche o da altri impianti già esistenti o in evidente stato di saturazione. A tal fine, il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati

che il commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto discariche ovunque vuole, si parla di aprire nuove discariche, di utilizzare le discariche autorizzate o realizzate dal commissario delegato e dal prefetto, praticamente ci facciamo fare prigionieri dal commissario con dei poteri straordinari che non ha mai avuto nessuno.

l'emendamento 5.2 della Commissione sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge. esprime la preoccupazione che andiamo ad insistere su discariche su cui c'era stato un impegno per la chiusura, come Ariano Irpino e Tufino, che sono nel testo del Governo, nel testo del decreto-legge che è giunto alla nostra approvazione. Con l'emendamento in discussione noi cancelliamo proprio la parte che preoccupa il senatore Matteoli, ma anche noi. Non c'è più Paenzano 2 nel Comune di Tufino, non c'è più Riconta nel Comune di Villaricca, non c'è più Difesa Grande nel Comune di Ariano Irpino. Se dovessimo ritirare l'emendamento 5.2, vivrebbe il comma

Presidente, comprendo lo spirito dell'intervento del relatore: vorrei però che l'eliminazione formale non restasse tale, ma fosse un'eliminazione sostanziale. ma fosse un'eliminazione sostanziale. Conoscendo la storia e tenendo presente, tra l'altro, che nell'articolo iniziale vi era una sorta di protezione per le discariche oggetto di provvedimenti giudiziari all'entrata in vigore del decreto ad oggi ci troviamo, nel caso di Difesa grande, nella condizione di un sequestro confermato in sede di riesame, a mio avviso questo elemento bisogna inserirlo e così facendo risolveremo il problema.

Presidente, mi rivolgo innanzitutto ai colleghi dell'opposizione e all'ex ministro Matteoli: chiedo di considerare con attenzione l'emendamento 5.2 che proponiamo come Commissione con il miglioramento che è intervenuto adesso in Aula grazie agli interventi del senatore Palumbo e del senatore Barbato. L'ex ministro Matteoli sa bene (ed è questo il punto delicato) che bisogna trovare, soprattutto nel caso dei rifiuti, soprattutto in una situazione così delicata come quella della Campania che è sotto gli occhi di tutti, un punto di equilibrio fra il rispetto delle sofferenze delle popolazioni che hanno già subito tantissimo (l'esempio della discarica di Villaricca è sicuramente calzante) e la necessità di affrontare l'emergenza nell'emergenza, che è quella con cui ci stiamo misurando in questi giorni. non mi sente - che stiamo affrontando un problema dell'emergenza nell'emergenza, proprio perché non si sono risolti i problemi strutturali in oltre 13 anni di commissariamento.

di quanto invece aveva inizialmente proposto il Governo - i nomi di tre discariche, alcune delle quali erano anche sottoposte a provvedimento di sequestro da parte della magistratura (quindi c'era un evidente conflitto). I tre nomi non esistono più; si dà mandato al commissario di trovare i luoghi dove smaltire i rifiuti, ma, contemporaneamente, gli si dice che che deve tener conto di quanto è successo nel passato e del fatto che ci sono alcuni Comuni della Campania che hanno sofferto più di altri e che, pertanto, deve stare particolarmente attento e cercare prioritariamente da altre parti gli eventuali posti. Questo mi sembra il punto di equilibrio più avanzato. Mi rivolgo anche ai colleghi che erano con noi in Commissione e che hanno studiato, credo con uno spirito molto costruttivo, questo provvedimento; mi rivolgo a loro per fargli capire che questo è il punto di equilibrio più avanzato possibile, che risolve, o almeno tenta di risolvere, l'emergenza nell'emergenza.

lui ha ricordato soltanto Difesa Grande, ma c'è anche il problema di Montesarchio, nella nostra Provincia di Benevento), suggerirei al relatore e al Governo di tenere in considerazione

fosse d'accordo la maggioranza (che invito ad essere attenta all'approvazione di questo emendamento), certamente avremmo risolto il problema che affligge la comunità campana, che è quello di intervenire su quelle già realizzate.

che le spese che saranno prodotte debbano far carico sul bilancio della Regione, che è l'unica vera responsabile del disastro della raccolta differenziata delle immondizie e dei rifiuti nella nostra Regione Campania.

"Il link apre una nuova finestra"). In relazione alla richiesta avanzata dal senatore Storace in apertura di seduta, il Presidente del Senato ha confermato quanto da lui già comunicato al Presidente della Commissione affari costituzionali in merito in merito alla applicazione in Commissione del comma 4 dell'articolo 78 del nostro Regolamento. La norma in questione riconosce certamente a ciascun senatore il diritto di avanzare proposte di deliberazione per parti separate anche relativamente a singole disposizioni del decreto legge o del disegno di legge di conversione. Diritto questo mai in alcun modo contestato e che può, pertanto, essere liberamente esercitato sia in Commissione che in Assemblea. Tuttavia, una volta riconosciuta l'esistenza di questo diritto, per la sua concreta applicazione non ci si può non rivolgere alle norme di carattere più generale che riguardano la votazione per parti separate, come indicate nel comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento. Tale comma prevede appunto che, una volta richiesta la votazione per parti separate, l'Assemblea deliberi sulla proposta per alzata di mano, senza discussione. Solo una volta accolta la proposta stessa, si potrà procedere alla votazione per parti separate. Cosa che, analogicamente, non può non applicarsi anche in Commissione. A conforto di questa decisione della Presidenza, si può ricordare un primo conforme precedente del 3 agosto 1994, nonché due precedenti conformi del 13 giugno e del 18 luglio 2006. Non sfugge senz'altro alla Presidenza che in tale ultima occasione il senatore Storace confermò la propria contrarietà: e la Presidenza ne prese atto. La Presidenza non ha però difficoltà a sottoporre anche questa questione all'attenzione dei colleghi Centaro e Zanda che, nella riunione della Giunta per il Regolamento del 26 ottobre scorso, hanno avuto mandato a riferire alla Giunta stessa sui quesiti regolamentari portati nei mesi scorsi all'attenzione dell'Assemblea. Onorevoli colleghi, comunico che, in relazione alle richieste avanzate questa mattina da vari Gruppi, la Presidenza ha acquisito la disponibilità del Governo a riferire domani all'Assemblea, alle ore 15, sulla situazione nei Territori Palestinesi. L'ordine del giorno della seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 15, è pertanto integrato con tale dibattito, nel quale i Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno e il Gruppo Misto Seguirà poi il sindacato ispettivo, come già previsto. Avverto, inoltre, che la seduta della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale,

Voglio apprezzare la tempestività, perché si è risposto ad una domanda che non avevo ancora posto in Senato, visto che quest'oggi ho semplicemente preannunciato la mia intenzione di porre una questione.

si dice, da parte degli Uffici della Presidenza del Senato, che ci sarà un' ulteriore approfondimento della questione. Se ci sarà tale ulteriore approfondimento, non si può agire in Commissione come se non ci fosse tale necessità di approfondimento. Cosa voglio dire, signor Presidente? Lo dico senza volontà polemica, perché credo che tutti abbiamo interesse - oggi governa uno domani governa un altro - ad evitare forzature. Lei, signor Presidente, ha fatto riferimento in questa nota, se non ho capito male, all'articolo 102, comma 5, del nostro Regolamento, il quale stabilisce una semplice regola sulla procedura nelle votazioni: cioè, se io sollevo una questione al fine di votare per parti separate, l'Assemblea decide per alzata di mano, senza discussione, su quella questione.

Mi riesce difficile immaginare che si possa adottare la stessa procedura persino, presidente Angius, sulle questioni legate all'esistenza dei presupposti di costituzionalità. Perché dico questo (e mi scuso se faccio perdere un minuto Esiste l'articolo 78 del nostro Regolamento, il quale dice che un decreto può essere esaminato interamente o per parti in relazione ai presupposti di necessità e urgenza,

da approfondire. Posso pregarla di evitare forzature in questa fase in Commissione? Altrimenti diventa difficile ragionare. Non voglio accusare il Presidente della Commissione, il cui garbo ho apprezzato in tantissime occasioni; oggi abbiamo avuto un momento di scontro e mi dispiace, perché non è mia volontà offendere alcuna persona. Ma dico: non c'è elemento di certezza che possa dire che l'articolo 102 prevale sul 78 perché, se fosse questa la ragione, mi deve dire, Presidente (questo è il quesito che pongo), in quale sede, Assemblea o Commissione affari costituzionali, un senatore ha il diritto di avanzare una proposta di stralcio rispetto all'inesistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. Mi spiego ancora meglio meglio (e lo dico al Segretario generale che ha compreso meglio di tutti noi): la proposta di votazione per parti separate precede la discussione sulla proposta. E se la discussione sulla proposta viene dopo, ma si vota per votazione per parti separate, per alzata di mano senza discussione, quella proposta non solo non sarà mai votata, ma nemmeno discussa. Ecco perché c'è da fare attenzione. Parliamo di procedure che riguardano l'articolo 77 della Costituzione, cioè norme entrate in vigore nel momento in cui un decreto viene al Senato. Ecco perché, Presidente, non è una questione che si può risolvere certamente nei cinque minuti di discussione che abbiamo qui.

perché uno dei precedenti ai quali ho fatto riferimento ha riguardato proprio me ed esattamente lei appunto il giorno 18 luglio 2006. Quindi, va benissimo.

non impedisce a nessuno di avanzare delle proposte di carattere procedurale, come già abbiamo detto; d'altra parte, ha la responsabilità di dare un'interpretazione del Regolamento e la dà. Contemporaneamente, però, affida a un supplemento di valutazione, come è stato detto nella risposta del Presidente, alla Giunta per il Regolamento. Quindi, la questione, da questo punto di vista, è trattata nel modo più possibilmente garantista per tutti.

affatto è il diritto di un senatore di chiedere votazioni per parti separate anche rispetto alla valutazione della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza che riguardino un provvedimento all'esame della Commissione affari costituzionali. Questo diritto è previsto, come dice giustamente il senatore Storace, nell'articolo 78 del Regolamento, il quale appunto prevede che anche la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione possa riguardare parti del provvedimento e, quindi, possa essere affidata ad una votazione per parti separate. Ma se l'articolo 78 è - diciamo così - la norma sostanziale, quella cioè che riguarda l'esistenza del diritto, altra è la norma procedurale, quella cioè che regola le modalità attraverso le quali questo diritto può essere esercitato. Qui, in assenza di una previsione esplicita che riguardi questo particolare esame e comunque, complessivamente, i lavori di ciascuna Commissione, si fa rinvio, ovviamente non esplicito, come sempre accade nell'interpretazione e nell'applicazione dei Regolamenti parlamentari, a quella norma del Regolamento che prevede la procedura perché questo diritto venga in essere. E la procedura è appunto quella, richiamata

ora mi importa, senatore Storace, sottolinearle che nessuno mette in discussione il diritto di chiedere che venga votata per parti separate la questione relativa alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.